Di chi sono le due schede a fianco della senatrice Rame?

Invito i colleghi a votare ciascuno dal proprio posto.

«Signor Presidente, come già ti avevo informato in mattinata, Ti confermo che la mia assenza dall'aula del Senato di questo pomeriggio è stata dovuta alla concomitanza della riunione della Commissione Mista Italia-Qatar che copresiedo, nella mia qualità di Ministro del Commercio Internazionale, assieme al mio omologo del Qatar dott. Yousuf Kamal, ministro delle Finanze e dell'Economia. La riunione, fissata da svariati mesi proprio per oggi 18 luglio, riveste carattere istituzionale e coinvolge, come tutte le Commissioni Miste di questo tipo, diversi Ministeri ed altre Amministrazioni, nonché alcune delle più importanti aziende dei due paesi su temi di mutuo interesse economico. Come sai, si tratta nel caso di specie di rilevantissimi interessi economici, inclusa la definizione della complessa questione riguardante il rigassificatore di Rovigo che, proprio nel quadro della Commissione Mista, ha trovato soluzione con reciproca soddisfazione. Inoltre, la riunione era stata rinviata già due volte e quindi mancare questo appuntamento sarebbe stato grave nei confronti dei nostri interlocutori. La folta delegazione del Qatar si trovava peraltro a Roma già da ieri, quando è stato calendarizzato il dibattito sulla legge comunitaria. un "Sottosegretario per le Politiche Europee", il governo è stato rappresentato in successione dai sottosegretari Li Gotti, Scotti e D'Andrea che ringrazio. Ti sarei grata di comunicare pertanto ai capigruppo ed ai colleghi senatori il mio rammarico per non aver potuto partecipare alla sessione pomeridiana del Senato per queste inderogabili ragioni di ufficio nella mia qualità di Ministro del Commercio Internazionale

Signor Presidente, intervengo solo per confermare e puntualizzare quanto scritto nella lettera, ivi compreso il fatto di avere avvertito la Presidenza e il presidente Marini di questa circostanza. Vorrei ringraziare i Vice ministri e i Sottosegretari che autorevolmente rappresentavano il Governo e sottolineare ai colleghi tutti l'importanza della riunione di ieri con i colleghi del Qatar, che immagino non vi sia sfuggita,

Confermo, altrettanto, che come Ministro delle politiche europee non ho un Sottosegretario. Mi auguro che i lavori di questa mattina, con la collaborazione di tutti, possano proseguire in modo soddisfacente.

relativamente al rapporto tra Governo e Senato della Repubblica e, specificatamente, tra il ministro Bonino, la nostra 14a Commissione e, più in generale, l'Aula.

con i colleghi di Governo del Qatar era già stata rinviata due volte. Forse, avremmo diritto di sapere per quali motivi di maggiore rilievo dell'essere presenti in Parlamento è stato possibile rinviare due volte quella riunione. In secondo luogo, è vero che il Ministro non dispone né di un Sottosegretario né di un Vice ministro per le politiche comunitarie, ma è vero anche che il Governo avrebbe potuto essere rappresentato

avendo manifestato ostilità nei confronti del Ministro su una questione e avendo ricevuto essa stessa ostilità politica da parte del Ministro su altra questione, ha fatto mancare due volte il numero legale.

*(UDC)*. Signor Presidente, prendo atto dell'importanza della riunione con il Ministro del Qatar per sostenere gli interessi della crescita economica del Paese e dell'interscambio tra i due Paesi: vorrei, però, segnalare al signor Ministro l'importanza della responsabilità che ella ha verso l'Aula parlamentare quando io sono abituato a pensare che il rapporto con il Parlamento abbia precedenza su qualunque altro e vorrei vorrei segnalare alla Presidenza che, in effetti, la legge comunitaria viene considerata come fattore di scarsa importanza da immettere nei momenti vuoti dell'attività parlamentare sono testimone io stesso - che il Ministro venga avvertito con grave ritardo della necessità della sua presenza in Aula. Questo non è un aspetto secondario. Lo dice il fatto che ancora non abbiamo assimilato la centralità ed importanza della politica europea. europea. Per questo, signor Ministro, devo ripeterle ciò che le ho detto ieri: non si può gestire la legge comunitaria come un adempimento burocratico, anche perché non si tratta solo della legge comunitaria, ma della relazione sulla partecipazione dell'Italia alle istituzioni europee ed è argomento di grandissimo rilievo politico perché tutte le grandi questioni della politica passano attraverso l'Europa. Signora Ministro, non le sfuggirà certo che la sua assenza in Aula

nel giorno successivo a quello in cui con una lettera lei segnala il suo forte dissenso rispetto ad una soluzione preconizzata in materia di pensioni. Tale materia la riguarda non solo perché riguarda tutti i Ministri, ma in quanto Ministro per le politiche comunitarie, perché essa viola un preciso impegno che il Governo italiano ha assunto in sede comunitaria. Ciò avviene nel momento in cui si propone una legge comunitaria che somiglia molto ad un autobus, nella quale la peculiarità della politica comunitaria viene dispersa dall'inserimento di molti elementi che non hanno qui il loro ruolo e il loro posto adeguato. Avviene nel momento in cui ci vengono avanzate alcune proposte da parte del Governo, sulle quali sono convinto che lei non può essere d'accordo, perché ripugnano non solo ad una liberista per convinzione come lei

e dalla difficoltà a rappresentare un Governo nel quale lei non si sente pienamente rappresentata e del quale, quindi, non si sente pienamente rappresentante. Credo che questi elementi politici non possano sfuggire all'attenzione dell'Assemblea. Non siamo qui a realizzare un adempimento burocratico, ma a parlare di politica europea. Mi auguro pertanto, signor Ministro, che lei esprima con chiarezza le linee di politica europea: quali non so, se le sue personali o quelle che sembrano prevalenti all'interno del Governo!

Dalla stampa abbiamo appreso una notizia grave e delicata: dopo mesi di vigenza del bando per il trasferimento della partecipazione di controllo pubblico in Alitalia,

queste sue osservazioni non hanno, insisto, una loro pertinenza. Può sviluppare le sue argomentazioni - preoccupate, mi sembra di capire e giustamente - a conclusione di questa seduta, quando mi riservo di darle la parola. FRUSCIO *(LNP)*. Pensavo che una preoccupazione che lei definisce giusta potesse interessare tutti noi. PRESIDENTE. Lo potrà fare, senatore Fruscio, anche con un margine di tempo più ampio di

Signor Presidente, da quando sto in Senato, cioè dal 1996*, l'iter* del disegno di legge comunitaria è stato sempre improntato ad un confronto mai conflittuale sotto il profilo delle diversità politiche di maggioranza e opposizione, perché finalizzato all'adeguamento del nostro sistema alle regole europee. non vi è stata mai una dinamica tipica di confronto d'Aula tra maggioranza e opposizione. Vi è stato sempre un confronto sereno, con un *iter* che si è sviluppato anche nell'arco di alcuni mesi, non soltanto di poche settimane, ma in cui tutto è stato improntato sempre a questa dinamica e a queste regole; che io ricordi, non ci sono eccezioni. Mi spiace dover rilevare

accade che in Aula ci si trova dinanzi ad un testo appesantito in Commissione da norme che introducono deleghe o che addirittura intervengono in maniera pesante su temi ambientali, senza essere state nemmeno esitate con un parere della Commissione industria o della Commissione ambiente. Quindi, troviamo introdotti in questo contenitore, che è stato sempre storicamente neutro e di ampia condivisione, temi invece di dibattito politico forte, che secondo me non andavano inseriti in questo contesto, ma in contesti tipici autonomi. Noi, ignari di questo fatto, signor Presidente, abbiamo accettato in Conferenza dei Capigruppo la piena e immediata calendarizzazione di questo provvedimento, ma le posso assicurare, e la prego di credermi, che personalmente, ove avessi avuto contezza di questo scenario, non lo avrei condiviso e mi sarei opposto alla calendarizzazione di questo tipo di testo, non votando il calendario per la prima volta in questa legislatura. Infatti, fino ad oggi, grazie anche alla mediazione del presidente Marini, abbiamo sempre votato all'unanimità le proposte della Presidenza.

Però, signor Presidente, mi permetto di fare appello alla Presidenza, al relatore e ai colleghi di maggioranza, di realizzare un momento di riflessione su quanto si sta consumando in questa Aula. Facciamo in modo di ricondurre il tutto al rispetto delle nostre regole comportamentali. Facciamo in modo che da questo testo vengano espunti temi che possono costituire oggetto di legislazione tipica di settore

ma le significo che, ove questo non dovesse succedere, naturalmente saremo costretti ad assumere atteggiamenti diversi che - la prego di credermi - non vorremmo assumere.

signor Ministro, lei non può venirci a dire qui che non è venuta in Aula perché stava lavorando, perché lavora tutti i giorni della settimana. Dire che non è venuta qui perché stava lavorando significa tacere due verità. La prima è la verità delle difficoltà con la sua maggioranza. In secondo luogo, Ministro, il fatto di venirci a dire che era impegnata con i rappresentanti del Qatar lo trovo anche un po' offensivo, perché lei è stata votata e rappresenta il popolo italiano e non il popolo del Qatar - glielo ricordo -, e il popolo italiano, nel momento della sovranità, si confronta qua.

se ne faccia imprestare qualcuno degli oltre cento che ci sono, magari qualcuno che cambi casacca e venga a aiutarla, per carità. Ripeto: la sovranità popolare si esercita in questo Parlamento. Presidente, lei non può dire: l'equivoco. Ma di quale equivoco stiamo parlando? Non siamo bambini nati ieri. Qui c'è una difficoltà politica da una parte, e c'è evidentemente un nodo istituzionale e anche di rispetto Non è possibile che in quest'Aula, Ministro, ieri sia successo che su argomenti molto importanti ci fosse un Sottosegretario che diceva

fare la formazione dell'Italia! Qui stiamo parlando di leggi, Ministro, che stanno mettendo in discussione i diritti dei cittadini nel campo della giustizia e in campo economico. Non possiamo lasciare una discussione così importante nelle mani, non dico dell'ultimo dei Sottosegretari, ma di un componente del Governo che non sa di cosa stiamo parlando. Allora, Ministro, lei non deve rivolgersi a noi, ma all'altra parte, perché ha avuto una fiducia a termine: il primo segnale lo ha già lanciato il Gruppo di Rifondazione

a meno che non ci sia una retromarcia su determinate posizioni. E questo, Ministro, è il nodo politico. Per quanto riguarda i contenuti, già ieri il presidente Castelli ha argomentato

molti di coloro che sono intervenuti, ieri il ministro Bonino non ha partecipato ad una seduta importante, ma questa mattina ha avuto la cortesia di spiegare con una lettera il motivo della sua assenza. Si può ritenere sufficiente o meno la spiegazione, ma il Ministro ha avuto la cortesia di giustificare la sua assenza di fronte all'Aula del Senato ed io ho apprezzato questo gesto del ministro Bonino. Veniamo ora all'argomento della nostra discussione.

se questo testo è firmato dal relatore, quindi non dalla Commissione, come sia possibile riprendere i nostri lavori senza che ci sia una riunione della Commissione che esamini tale nuovo testo e, soprattutto, come sia possibile riprendere i nostri lavori senza che sia dato un tempo sufficiente per poter presentare eventuali subemendamenti. A me pare che sia arrivato il momento di dover decidere questo; non possiamo continuare i nostri lavori. Se non avessi ricevuto questo testo o se si smentisse

convocare la Commissione e dare ai Gruppi un tempo sufficiente per poter esaminare la possibilità di presentare subemendamenti. *(Applausi

il presidente Matteoli - che c'è stato un atto di cortesia del Ministro, che è avvenuto, lo ricordo al presidente Matteoli, non questa mattina, ma ieri sera, quando è pervenuta quella lettera al Presidente del Senato. Alla Presidenza del Senato non sfuggono - questo lo dico ai colleghi Stracquadanio, Vegas, Buttiglione, Fruscio, Schifani, Polledri e allo stesso Matteoli - gli gli elementi di difficoltà politica che sono andati emergendo nella discussione della legge comunitaria e che sono, più in generale, all'attenzione del Governo e della maggioranza in relazione alla discussione e al confronto che c'è, interno al Governo e alla maggioranza, in riferimento ad altri provvedimenti che il Governo si accinge a varare. Sono davanti agli occhi di tutti e quindi sono ben noti. Tuttavia, devo dire ai colleghi che sono intervenuti che, in relazione all'episodio che abbiamo vissuto ieri, come dice la lettera stessa, si è trattato effettivamente di un equivoco spiacevole. Infatti, ci ricorda il Ministro, all'inizio della lettera indirizzata al Presidente del Senato: «Signor Presidente, come già ti avevo informato in mattinata, Ti confermo che la mia assenza dall'aula del Senato di questo pomeriggio è stata dovuta alla concomitanza della riunione della Commissione Penso si sia trattato di uno spiacevole equivoco che, tra l'altro, se non ci fosse stato, avrebbe consentito nella giornata di ieri una discussione generale su altri provvedimenti e così, invece, ci troveremo la prossima settimana con una difficoltà rispetto al calendario per concludere nei tempi che avevamo prefissato i nostri lavori prima della pausa estiva.

non possa permanere un'opinione contraria al provvedimento o a suoi singoli aspetti, che può essere del tutto legittimamente confermata in quest'Aula e ribadita con il voto conseguente.

l'assoluta asimmetria, l'assoluta azione farisaica e l'assoluto imbroglio della politica internazionale, in relazione alla questione degli armamenti nucleari,

la gravissima tensione succeduta nel 1962 per i missili a Cuba. Il Trattato è stato ratificato poi nel 1970, quando ha raggiunto un numero sufficiente di Paesi firmatari e da allora l'AIA, l'agenzia che controlla questo trattato dell'ONU, ha diviso il mondo in Paesi possessori e non possessori di armi nucleari. Dico subito ‑ anche perché sono abituato a vedere prima le cose positive ‑ che il Trattato ha dato dei frutti immediati: il Sudafrica ha distrutto i suoi armamenti nucleari, mentre il Brasile e l'Argentina, che erano avviati su quella strada, hanno rinunciato. Il Trattato è stato molto utile per l'implosione dell'Unione Sovietica, quando i Paesi dell'Est dell'ex Unione Sovietica si ritrovarono con armamenti nucleari, che appunto il Trattato e la collaborazione con le organizzazioni internazionali permisero di mettere di mettere in sicurezza. Voglio anche ricordare, però, che alcuni Paesi, quali l'India e il Pakistan, si sono dotati successivamente di armamenti nucleari,

per la Corea del Nord, che comunque ha due testate, mentre anche il Giappone, nonostante la tragedia di Nagasaki e Hiroshima del 9 e 6 agosto 1946, pare intenzionato ad andare in questa direzione. Colleghi, poiché stiamo parlando di sanzioni all'Iran, vorrei ricordarvi la situazione attuale sul pianeta per le testate nucleari: nucleari: gli Stati Uniti hanno 10.280 testate, la Russia 8.459, la Gran Bretagna 200, la Francia 390, la Cina 420, l'India 95, il Pakistan 90, Israele 200 e la Corea del Nord

di "Stone Ax". Vengo al dunque: di fronte a questa situazione, possiamo continuare a fare gli ipocriti; possiamo continuare a dire che non vogliamo gli sviluppi nucleari e ignorare che il Trattato di non proliferazione nucleare non solo impedisce nuove acquisizioni di nucleare militare, ma obbliga i firmatari anche alla riduzione dei propri armamenti e che l'Italia, che in tal senso ha svolto da sempre un ruolo positivo, ha sottoscritto un impegno alla denuclearizzazione del proprio territorio,

Nobel: fino a quando alcuni tra noi sceglieranno di mantenere arsenali nucleari, questi continueranno ad essere attraenti anche agli altri; se vogliamo evitare l'autodistruzione, le armi nucleari devono smettere di far parte della nostra e non avere ruolo nelle nostre strategie di sicurezza. A questo fine, dobbiamo assicurarci che nessun Paese acquisisca queste terribili armi e lavorare perché gli Stati che hanno il nucleare facciano passi concreti per il disarmo. Israele con 200 testate e il povero Mordechai Vanunu, il tecnico israeliano che aveva denunciato la base di Dimona, è di nuovo sei mesi in galera dopo esservi stato 18 anni; abbiamo il Trattato a seconda della geopolitica degli interessi dell'impero: quali ipocrisie vogliamo continuare a fare

coscienza: così non si può andare avanti, perché il mondo non ci crederà; non ci crede quando chiediamo i diritti e non ci crede perché abbiamo una doppia bilancia e la bilancia è quella per cui quando Musharraf era nemico degli Stati Uniti era giustamente un criminale golpista

Non possiamo continuare a fare finta di essere giusti, di essere eguali e di trattare tutti secondo le nostre astratte caratteristiche quando poi, nel concreto, i giudizi sulle questioni vanno sempre riferiti solo alla alla nostra convenienza. O questo finisce o noi assisteremo all'autodistruzione non solo per il nucleare, ma perché gli altri popoli del mondo non ci crederanno più: non crederanno che le 200 testate di Israele sono legittime e la proposta della Lega Araba di denuclearizzare il Medio Oriente non viene accolta perché

A chi mi chiede di ritirare l'emendamento 28.100 dico che capisco (io poi sono più prodiano di Prodi), però vorrei ricordare che Prodi quando venne qui disse che sui problemi etici c'è libertà di coscienza e sicuramente i problemi etici non sono solo il controllo del corpo delle donne, degli stili di vita delle persone, degli embrioni e quant'altro, ma sono prima di alla pace. Sarei quindi in pieno diritto, secondo le parole di Prodi, di dissentire anche da questo Governo per la mia coscienza individuale; ma siccome sono più prodiano di Prodi, propongo al relatore e al Governo di ritirare l'emendamento 28.100 presentando in sostituzione un ordine del giorno che, se il Presidente mi da tempo, vado a leggere.

che hanno posto una questione su come procedere nei nostri lavori della determinazione della Presidenza, che sarebbe la seguente: continuare nell'esame degli emendamenti e degli articoli non accantonati sino ad arrivare a discuterli ed approvarli, in modo tale da esaurire questa parte della nostra discussione. Una volta arrivati agli articoli che sono stati accantonati,

e per altri che potrei esporre poi in dichiarazione di voto, se non dovesse essere disposto l'accantonamento dell'articolo 28, faccio mio l'emendamento del senatore Silvestri.

è un po' un lavarsi la coscienza a buon mercato. I colleghi della sinistra, infatti, i pacifisti, molto attenti a queste tematiche, avrebbero dovuto leggere con attenzione la relazione annuale che il Governo

ed è giusto limitare e controllare i traffici che avvengono verso questi Stati - dovremmo guardare, innanzitutto, in casa nostra. A leggere la relazione, sembra che il primo Stato canaglia sia l'Italia che, dopo avere firmato un'infinità di protocolli, si permette

parere contrario. Voglio solo ricordare, al di là del merito, che forse necessita di altro tipo di dibattito in altra sede per i rilievi posti, che in questa fase si tratta di dare applicazione

del 2006. Lo dico solo per informazione di tutti. Nel merito, in altra sede può riaprirsi un dibattito. Per questo il parere del Governo è contrario.

solo una precisazione: il senatore Silvestri nel suo intervento si è detto disponibile a ritirare il suo emendamento a condizione che da parte del relatore e del Governo ci sia la disponibilità ad accogliere un ordine del giorno. Ebbene, in merito non è arrivata alcuna risposta. Il Governo e il relatore comprenderanno che, essendo stato fatto proprio dall'opposizione, se non vi è l'accettazione dell'ordine del giorno esistono un po' di problemi di coerenza.

non si presti il doveroso omaggio ad un italiano del quale oggi ricorre il quindicesimo anniversario della tragica scomparsa. Mi riferisco a Paolo Borsellino e ai ragazzi che provvedevano alla sua tutela e che sono morti con lui in quel terribile pomeriggio di domenica. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in questa circostanza è facile scadere nella retorica e ogni parola suona stucchevole, per cui mi fermo qui. ricordare che, come il più efficace elogio del giudice è stato quello scritto da un avvocato (e che avvocato!), così non trovo parole più adeguate per ricordare in estrema sintesi un magistrato come Paolo Borsellino di quelle adoperate da un delinquente che ebbe a che fare con lui. Non ne menziono il nome, non importa, ma è sufficiente dire che è stato uno dei primissimi e non fasulli collaboratori di giustizia, convinto da Borsellino a rompere con Cosa Nostra prima che entrasse in vigore la legge che riconosceva benefici e sconti di pena, tutela e così via. via. Questo primissimo collaboratore di giustizia affermava di aver scelto di rompere con l'ambiente di provenienza perché aveva individuato in Paolo Borsellino un autentico uomo d'onore, uomo d'onore, ma non come la mafia intende questa espressione, bensì come un siciliano e italiano autentico, quale era Borsellino, assume in fino in fondo la propria responsabilità. Lo è stato realmente sino in fondo e lo ha fatto perché un giorno ha assunto un impegno d'onore nei confronti della propria comunità e della propria Patria, che ha pagato nel modo in cui tutti sappiamo. Ecco, Presidente, credo che quest'Aula all'onore di Paolo Borsellino, al suo sacrificio e a quello degli uomini addetti alla sua scorta debba rendere oggi, nelle modalità che lei riterrà più opportune, l'omaggio più doveroso.

ho due ricordi personali dai quali vorrei partire. Il primo risale al 20 luglio del 1988, Paolo Borsellino denunciò la solitudine nella quale Giovanni Falcone si trovava a condurre il proprio lavoro, la crisi e la dissoluzione del *pool* antimafia di Palermo. Egli fu convocato davanti al Consiglio superiore della magistratura per rendere ragione di queste gravi accuse rivolte a chi aveva la responsabilità di guidare allora l'ufficio istruzione presso il tribunale di Palermo e ci raccontò come il *pool* antimafia era stato messo in condizione di non poter continuare il suo proficuo lavoro. Nell'ira sincera che Paolo Borsellino manifestava allora davanti al Consiglio superiore della magistratura vi fu anche un riferimento che è rimasto impresso nella mia memoria. Egli affermò: nell'estate dal 1985 lo Stato non era in grado di garantire l'incolumità mia, quella di Giovanni Falcone e quella degli altri magistrati del *pool*, per cui dovemmo andare a scrivere l'ordinanza‑sentenza del maxiprocesso all'Asinara. Abbiamo lavorato lì perché non potevamo stare a Palermo quando sono tornato - ci disse Paolo Borsellino - lo Stato mi ha mandato un documento, un pezzo di carta: si trattava della fattura che ho dovuto pagare per il mio soggiorno all'Asinara. noi che lo ascoltavamo eravamo con gli occhi aperti, incapaci di dargli un un sostegno che andasse al di là delle parole, nella battaglia che qualcuno di noi ha condotto per sostenere il *pool* antimafia. Il secondo ricordo personale

Paolo perché non fai domanda e torni anche tu a lavorare qui? Vedrai che al CSM si formerà una maggioranza per il tuo ritorno a Palermo. E lui, aveva una sigaretta tra le dita come sempre, o quasi sempre, mi rispose: «Ma tu credi davvero che questi possano tollerare che Falcone ed io lavoriamo insieme nella Procura di Palermo? Non lo tollereranno mai!». Infatti, mai è avvenuto che essi lavorassero assieme in quell'ufficio. Nessuna retorica, dunque, ma soltanto il ricordo di persone che hanno combattuto per la Costituzione repubblicana, per la legalità, per la legalità, contro la mafia, senza guardare in faccia nessuno, senza piegarsi, di idee politiche diverse (perché Falcone e Borsellino avevano idee politiche diverse

non capivano il senso dell'impegno di uomini che hanno le loro idee (perché anche i magistrati hanno le loro idee ed opinioni, anche di parte) ma che, se sono grandi magistrati, non si fanno guidare da quelle opinioni ma soltanto dalla lealtà nei confronti della Costituzione e dello Stato democratico. È la stessa lealtà degli uomini della scorta e di Emanuela Loi, la donna poliziotto che aveva scelto di stare vicino a Paolo Borsellino, e che sono morti con Falcone e Borsellino per difendere la dignità dello Stato. Essi erano e rimangono nella nostra memoria come servitori della patria ed eroi della Costituzione repubblicana. Noi li ricordiamo così, insieme, e cerchiamo,

commemorarlo e in questi anni ho dovuto commemorarlo abbastanza spesso. Ricordo solo che, insieme a Paolo, abbiamo dovuto commemorare Giovanni Falcone. Subito dopo, toccò a me, da solo, commemorare Borsellino. Per me Paolo è stato un fratello, con il quale ho condiviso tanti anni di lavoro e con il quale ho combattuto tante battaglie. Lo ricordo proprio per quel suo impegno come vero uomo delle istituzioni. Ho scritto una volta, commemorandolo su un giornale, che egli è stato un eroe borghese,

al mondo siciliano, nel senso di essere giudice al di sopra delle parti, e il suo essere anche amico,

quando il presidente Schifani ha prima ricordato in Aula che il presidente Marini oggi rappresenta noi tutti, oltre che l'intero Paese, alla commemorazione di Paolo Borsellino a Palermo, mi è sembrato giusto attirare l'attenzione sulla necessità, che anche noi abbiamo, di dedicare oggi il nostro ricordo a Paolo Borsellino affinché questo possa aiutarci a riflettere meglio sui nostri doveri rispetto ai temi della giustizia e, più ampiamente, della legalità del nostro Paese. Paolo Borsellino rappresentava e rappresenta nella nostra memoria - credo - nel cuore di tutti gli italiani, insieme con Giovanni Falcone, l'emblema, il simbolo della legalità; la legalità a tutti costi, la legalità al di sopra di tutto, la legalità sostenuta da una chiarezza, una trasparenza e un'onestà di pensiero che ha sempre guidato la loro azione. Ho avuto la fortuna di conoscere Giovanni Falcone, meno Paolo Borsellino, ma penso sia irrilevante. Tutti gli italiani conoscono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino; forse pochi italiani ricordano come la loro azione fosse spesso poco compresa, non condivisa, e non per motivi ideologici, da quella parte di magistratura che anteponeva l'appartenenza ideologica alla sostanza dei fatti, perché la loro limpidezza era evidentemente imbarazzante per tutti, per le coscienze di quei magistrati che, invece, a Palermo riempirono di veleni la vita e resero difficile l'operato di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino. Mi ha colpito molto il titolo di apertura di una *fiction* che la nostra TV pubblica manda in onda, che recita così: in un altro Paese, il lavoro di questi uomini sarebbe diventato esempio e memoria perenne per tutti e invece tante volte, troppe volte, il lavoro di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino è stato addirittura fatto oggetto di dileggio. Ricordiamo tutti quando, dopo l'attentato dell'Addaura, subìto da Giovanni Falcone, qualcuno ne mise addirittura in discussione la veridicità; qualcuno arrivò persino a sostenere che Falcone si era messo da solo quella bomba! Ecco, erano i veleni di un sistema giudiziario, talvolta appesantito da fardelli che noi riduciamo ad una parola, che spesso invochiamo e che raramente pratichiamo, quell'indipendenza della magistratura che, quando è esempio per tutti noi, lezione morale per tutti noi e garanzia certa della nostra democrazia e della nostra Costituzione. Grazie, Presidente, per averci consentito questi minuti di ricordo e di memoria di due uomini che restano un esempio per la magistratura tutta e per tutti noi cittadini italiani.

ci sono elementi oscuri che la precedente sentenza di condanna dichiara espressamente aperti; sono iniziate nuove indagini da parte della magistratura di Caltanissetta: ogni sforzo, dunque, deve essere compiuto perché sia fatta chiarezza fino in fondo sulle ragioni di quella strage e perché sia fugato ogni residuo dubbio. Chiedo in particolare al ministro Mastella, nel momento in cui la magistratura di Caltanissetta segnala difficoltà di organico e di mezzi per approfondire queste delicate indagini, che il Governo faccia interamente la sua parte per rendere possibile questo accertamento. L'Italia intera lo deve a Paolo Borsellino e ai servitori dello Stato morti con lui.

non può farci dimenticare, dietro parole di circostanza, alcune verità politiche e storiche di quegli anni che vivono ancora adesso.

voglio solo ricordare due aspetti. Il primo è che le peggiori campagne di accuse infamanti nei confronti del dottor Falcone e, di conseguenza, anche del dottor Borsellino non vennero soltanto dall'interno di certa parte della magistratura, ma anche da parte di esponenti politici di primissimo piano, di quella che fu chiamata, millantando, la "Primavera di Palermo",

Ci sta accomunando il ricordo di persone che hanno davvero illustrato al meglio la storia del nostro Paese.

Pregherei non solo lei, ma tutti noi, di bandire in questa circostanza qualsiasi pensiero che ci rimane, di giudizio o di valutazione politica,

il dottor Falcone di nascondere i segreti nei cassetti. L'ho negli occhi, come ho negli occhi le immagini della strage di Capaci. Non posso allontanare questi due ricordi, così come non posso fare a meno di constatare, Presidente, e concludo, che dopo Falcone e Borsellino è iniziata una stagione devastante per la nostra giustizia, che ha portato all'affermarsi di quello che loro non volevano e cui avevano fatto fronte in ogni caso, cioè il dominio del pentitismo, organizzato dai medesimi pentiti, contro la verità e contro la giustizia. Ciò ha portato a una fase buia nel nostro Paese, dove - grazie a Dio - la vita ha consentito che alcuni nostri colleghi

Presidente, onestamente avrei preferito che il ricordo di Borsellino fosse oggetto di una seduta speciale del Senato, nella quale si potesse intervenire non casualmente e in modo molto più

Signor Presidente, mi scusi, ma non credo che lei possa imporre il contenuto degli interventi ai colleghi. Detto questo, mi atterrò per quanto possibile - ad un atteggiamento sobrio, pur dicendo che la verità su questa vicenda va ancora tutta riscritta.

forse anche diversa sugli avvenimenti di allora. Presidente, colleghi, chi ha la ventura di salire lo scalone d'onore del Ministero della giustizia può vedere una targa di bronzo che commemora il decennale della morte di Giovanni Falcone. I casi della vita e la cronaca mi hanno portato ad avere l'onore di essere stato il Ministro *pro tempore* a porre quella targa ad imperitura memoria di Falcone, ma, evidentemente, anche di Borsellino, perché non si può mai parlare dell'uno senza ricordare l'altro. Furono accomunati nella vita e, purtroppo, anche nella loro tragica scomparsa. Ricordo - altro fatto eccezionale - che per la prima volta, in quella commemorazione, un Presidente della Repubblica varcò i cancelli di via Arenula e che nella mia prolusione posi una domanda, ovviamente retorica: furono Falcone e Borsellino eroi del nostro tempo? Sicuramente lo furono, tanto più - com'è stato ricordato prima dal collega Di Lello Finuoli - che non furono eroi per per una sorta di *Sturm* *und* *Drang* e per un impeto istintivo. No, loro sapevano perfettamente, a livello razionale, che sarebbero andati a morire e non hanno mai smesso un momento di

Allora, forse, ha ragione Bertolt Brecht: mai, come in questo momento, la sua frase «beato il Paese che non ha bisogno di eroi » risuona di fronte a noi.

Purtroppo, l'atmosfera per lui all'interno della magistratura si era fatta irrespirabile. Mi piace ricordare che fu un Ministro laico - come Martelli e come me - ad accoglierlo al Ministero della giustizia.

ringraziarla per il richiamo che lei ha fatto poc'anzi: di fronte a questi momenti ufficiali e di alto spessore la polemica politica dovrebbe essere messa da parte.

si unisce al ricordo di una delle vittime più illustri della guerra di mafia, quella guerra che in tanti, da vent'anni, combattono contro una piaga che noi siciliani ci portiamo dietro da un secolo. Oggi a Palermo si tengono tante manifestazioni, alcune delle quali anche *bipartisan*. Mi permetto di fare riflettere il il Parlamento, l'Aula del Senato sul fatto che c'è tanta stanchezza nei siciliani per questo continuo commemorare, se poi lo Stato - e con esso la politica - non riesce a sradicare in maniera definitiva la mala pianta della mafia. Credo che l'occasione di oggi di oggi e le iniziative anche forti che il Senato della Repubblica può intraprendere nel prossimo futuro debbano servire per invertire tutti insieme una rotta che fino ad oggi ci ha portato a fare barricate da una parte o dall'altra, ma che alla fine porta a vincere un fenomeno che rende noi siciliani sempre più indietro rispetto al resto d'Italia.

Mi sembra che abbiamo già operato una rottura rispetto alla discussione che stavamo svolgendo, dato il rilievo della questione sollevata giustamente dal senatore Mantovano, che ringrazio, però non possiamo affrontare un dibattito né sulla lotta alla mafia, né sui caduti per mano della mafia. È una giornata del tutto particolare, nella quale siamo rappresentati a Palermo dal presidente Marini. Tutto il Senato è rappresentato; quindi, mi atterrei a questo criterio. Chiedo scusa ai colleghi, ma in altra occasione e circostanza avranno modo di prendere la parola per esprimere il loro personale ricordo del

un grande servitore dello Stato, che proprio quindici anni fa fu barbaramente assassinato da mano mafiosa e criminale. Un servitore che ha posto al centro della sua azione di magistrato il prevalere della legalità, l'affermazione di ogni azione funzionale ad abbattere tutte le mafie. Borsellino è morto sereno per avere compiuto fino in fondo il suo dovere, per avere compiuto un'azione di disinquinamento sociale in una Regione dove la malapianta della mafia aveva corroso e continua a corrodere i pilastri di una civile convivenza. Noi oggi lo ricordiamo con sobrietà, con l'auspicio, espresso dal presidente Salvi, che la magistratura di Caltanissetta faccia piena luce sui mandanti di questo barbaro assassinio, rimuovendo tutti gli steccati che hanno impedito fino ad ora il conseguimento della verità. Auspichiamo, infine, che il Presidente del Senato voglia realizzare, nell'ambito delle iniziative annuali, una giornata per le vittime della mafia.

Io non ho avuto la fortuna di lavorare con Borsellino, ma credo che ogni magistrato avrebbe dovuto fare un'esperienza, sia pure virtuale, con questi due eroi della magistratura.

un rapporto abbastanza costante per un certo periodo di tempo con Borsellino, poco prima della sua morte, raccogliendo quegli stimoli e quelle iniziative che con la sua esperienza, e dopo la morte di Falcone, egli cercava di dare e dava costantemente al Ministero della giustizia. Quanto al fatto che costituisca e abbia costituito un esempio costante per la magistratura, debbo soltanto ricordare, dire o annunziare che nell'aula delle riunioni dell'Associazione nazionale magistrati campeggia una grossa fotografia di Falcone e Borsellino con la seguente scritta: al ricordo costante di come tutti i magistrati debbano poter dare il proprio impegno a difesa dello Stato e della legalità, quali che siano le loro idee. In questa prospettiva e con questo sentimento, rivolgo un pensiero affettuoso, ringraziando il Senato a nome del Governo per questa unità di emozione e di commozione, al ricordo di Paolo Borsellino. Desidero ringraziare tutti i colleghi che sono intervenuti con accenti sentiti e partecipati

riflessioni e pensieri che investono la storia del nostro Paese. Troppo spesso, nell'andare con la memoria alle vicende del passato, siamo portati, forse rispetto anche ad altri Paesi, a ricordare il peggio, e il peggio, nella storia anche della nostra democrazia recente, c'è stato. Abbiamo vissuto stagioni orribili che hanno scosso coscienze, distrutto famiglie, tolto all'Italia alcune delle sue menti, dei suoi uomini e delle sue donne più prestigiosi. Non ho conosciuto Paolo Borsellino, ma in una circostanza conobbi Giovanni Falcone; era una tarda primavera, a Palermo, e Gerardo Chiaromonte, allora presidente della Commissione Antimafia, mi disse: «Debbo incontrare Giovanni Falcone, vieni anche tu». Ci incontrammo a casa di un comune amico, per raggiungere la quale dovemmo fare mille peripezie - per ragioni di sicurezza, mi si disse -: cambiamenti di macchina,

anche perché avevamo alle spalle dei terribili delitti di mafia. Ad un certo momento, nel corso della cena, con una serenità disarmante disse, usando una parola diversa da quella che ha utilizzato poco fa il collega Di Lello: «È arrivata la polvere, molta». Lì per lì, appena pronunciata la parola non capii; ma subito dopo capimmo. Lo disse con una serenità e con una tranquillità non fatale, ma direi con la sicurezza rispetto a ciò che poi sarebbe avvenuto. Proseguimmo la cena: era sereno, tranquillo e distaccato. Lì capii - ma lo capii anche quando il suo amico fraterno, Paolo Borsellino, saltò in aria in via D'Amelio con i giovani ragazzi e ragazze della sua scorta che cosa vuol dire essere servitori dello Stato, che cosa vuol dire avere un'etica del dovere, che forse in questo nostro Paese abbiamo smarrito e il cui recupero io sento necessario e urgente. Queste nostre rievocazioni, questi nostri ricordi hanno un senso se quell'etica del dovere noi la consideriamo per tutti noi, soprattutto nell'esercizio pubblico delle nostre funzioni, il dono più prezioso che Paolo Borsellino, Giovanni Falcone e tutte le vittime della mafia ci hanno lasciato. *(Applausi dei dell'Italia civile e democratica alla quale noi, la nostra libertà e la nostra democrazia devono tanto, anzi forse devono tutto.

Signor Presidente, ho già illustrato la questione motivando la proposta di non passaggio agli articoli, che ora vorrei precisare meglio. Intanto devo correggere il senatore Sinisi, che ieri ha fatto un discorso

significa: tutte le pratiche che vengono fatte all'interno delle aziende private domani cadranno - non uso il condizionale perché anche noi siamo d'accordo, l'abbiamo approvata anche noi quella decisione quadro

se non semplicemente che il Governo è delegato a scrivere questa legge. Mi domando come il presidente Napolitano possa firmare un testo del genere. Ci avete abituato a tutto in questa legislatura e probabilmente passerà anche questo, ma credo che chiunque si astragga un momento dalla necessità di dover approvare l'operato del Governo possa capire che siamo veramente al di fuori di qualsiasi regola di di legislazione coerente. Non so più cosa dire, ormai ne stiamo vedendo di ogni colore in quest'Aula, vediamo anche questo. Presidente Salvi, mi appello a lei, a questo punto.

Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC ha votato contro la proposta di non passaggio agli articoli motivata con una ostilità generale generale alle modalità previste dalla legge per la equiparazione fra decisioni comuni e direttive. L'argomentazione testé svolta dal senatore Castelli però attira l'attenzione su di un altro aspetto, che non è di ostilità in generale, bensì di contenuto: è ovvio che questioni che riguardano la libertà dei cittadini meritano un'attenzione del tutto particolare.

Come ho detto nel mio precedente intervento, su temi del genere è necessario un confronto più attento e approfondito, mentre in questo caso ci troviamo a svolgere un dibattito affrettato ed inadeguato. Aggiungo che la legge consente anche fuori dalla Comunità di attivare modalità specifiche qualora se ne ravvisi l'opportunità. Vorrei invitare la signora Ministro a riflettere sulla opportunità di scegliere un canale differente

per cercare il modo, in una prossima legge comunitaria preceduta da adeguato confronto in Commissione o con apposito provvedimento legislativo, di affrontare con delicatezza adeguata al tema un problema che è stato preso in questa occasione troppo sotto gamba. Colgo l'occasione per ricordare che anche in altri punti di questo disegno di legge rileviamo

io ho lavorato su un disegno di legge che constava di 22 articoli e oggi sappiamo che gli articoli sono quasi 40. Una cosa

del confronto in Commissione, che poi è il modo in cui si esprime il vincolo parlamentare in questi casi specifici. Il Gruppo dell'UDC voterà a favore della proposta del senatore Castelli. *(Applausi del senatore Possa).*

Signor Presidente, a differenza di quanto pensano e dicono il senatore Castelli ed il senatore Buttiglione, la questione è stata molto approfonditamente affrontata all'interno della Commissione giustizia di questo Senato, non come Sottocommissione pareri, ma nel *plenum* della Commissione, e di questa tematica si è discusso in più sedute con particolare riferimento - tengo a dirlo - alla decisione quadro del 2003 relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato. avanzate diverse proposte di emendamenti, ci sono stati diversi punti in discussione - alcuni ne ricorderò - e sono intervenute decisioni della Commissione giustizia del Senato che hanno motivato nel contenuto in particolare la reiezione di alcune proposte, che erano arrivate alla Commissione, addirittura attraverso alcuni senatori, dall'Associazione delle banche. Per quanto riguarda la decisione quadro del 2003 sulla corruzione nel settore privato, è stato anche ricordato all'interno della Commissione giustizia come quella di riferimento sia una normativa che ormai è stata rappresentata a livello internazionale anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Anche per quanto riguarda le ulteriori decisioni quadro, alle quali si fa riferimento nel Capo III, si è svolta una specifica discussione su richiesta di senatori dell'opposizione,

c'è stata una dettagliata discussione proprio in relazione al concetto di sanzioni pecuniarie e a proposte emendative formulate sia da me che dal relatore della 14a Commissione, per integrare il testo della delega affidata al Governo. Quindi, dalla prima decisione quadro sulla corruzione nel settore privato all'ultima, che riguarda le sanzioni pecuniarie, le discussioni sono state ampie e dettagliate per chi era presente in Commissione e per chi voleva sentire.

di delegare il Governo ad inserire norme in materia, all'interno del codice civile o del codice penale. L'indicazione fornita dalla 14a Commissione, competente nel merito, è quella che risulta dal testo e anche la Commissione giustizia si era pronunciata in quel senso.

luogo la determinazione della collocazione sistematica nel codice penale, tant'è vero che si modificò l'indicazione contenuta nel testo del Governo al codice civile. i soggetti che possono essere autori di tale reato, la determinazione della fattispecie specifica, con tutte le sue modalità attuative e la finalità. in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali; Quindi, la discussione sia nella prima sede sia nell'altra è stata molto ampia, e non è vero che vi sia una delega in bianco al Governo, anzi, i criteri di delega sono estremamente stretti e direi abbastanza convincenti convincenti rispetto ad una delineazione di fattispecie, secondo il principio di certezza e di tipicizzazione tipica del codice penale. do atto al sottosegretario Scotti della riunione a cui ho partecipato, in cui ho difeso, come ho fatto anche in quest'Aula, il principio dell'equiparazione tra decisioni quadro e direttive e direttive che è contenuto nella legge e che comunque rappresenta la direzione verso cui si avvia l'ordinamento comunitario. Do anche atto che c'è stato da parte mia un equivoco: il cambiamento della numerazione ha indotto alcuni colleghi a segnalarmi il non passaggio in Commissione di un tema che invece in Commissione è passato. Mantengo tuttavia il giudizio di merito per cui, in questo caso specifico, i criteri di delega appaiono essere troppo vaghi e imprecisi e, data l'importanza della questione, sarebbe opportuno un esame più attento. Tengo a distinguere due prospettive: noi abbiamo votato contro il non passaggio agli articoli perché riteniamo che decisioni quadro e direttive siano giustamente equiparate; in questo caso specifico, non siamo convinti della soluzione che è stata adottata.

non riguarda solo la violazione degli obblighi inerenti all'ufficio, come era nel testo originario, ma un indebito vantaggio di qualsiasi genere, quindi è una previsione molto estensiva che dà una discrezionalità a mio avviso eccessiva. Tra l'altro, essa non riguarda solo i dirigenti che hanno deciso questo tipo di azione, ma qualsiasi lavoratore, per qualsiasi lavoratore coinvolto nel processo produttivo, anche l'operaio che trasporta il pacco, può essere imputato di questo reato, il che francamente mi sembra che vada un po' *ultra*. In questo senso,

che, pur restando nell'ambito della decisione quadro, forse va valutata meglio dal Parlamento nazionale. Si tratta infatti di diritti delle persone, di norme del codice penale, di fattispecie molto delicate che in questa sede sono state risolte in un modo, quanto formalmente ineccepibile, forse un po' troppo frettoloso e con una valutazione troppo estensiva della fattispecie penale, e sappiamo che estendere troppo le fattispecie penali è uno sbaglio da un punto di vista generale.

soppressivo delle medesime lettere, in modo da consentire poi una successiva valutazione nella sede di merito. le chiedo l'accantonamento dell'articolo 31 perché la peculiarità della materia impone a mio avviso una riflessione ulteriore.

al relatore, che in Commissione si è occupato della materia) una più puntuale tipicizzazione delle condotte eventualmente censurabili. Per fare ciò occorre del tempo. Quindi, se fosse possibile l'accantonamento lavoreremmo meglio per realizzare un obiettivo più coerente con le esigenze generali.

Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori perché proprio raffrontando i testi

Teniamo presente che la norma, sia nell'una che nell'altra versione, tenderebbe ad attuare una decisione comunitaria contro la corruzione nel settore privato. privato. Presidente, se così è e poiché le due ipotesi sono molto diverse, vorrei ricordare ai colleghi che l'ipotesi del testo originario riguarda una fattispecie criminosa prevista nell'ambito del codice civile per chi è titolare di funzioni particolari (direttori, amministratori, sindaci ed altre figure). Essa è giustamente collocata nel codice civile e in quel contesto vengono previste le sanzioni penali. l'ipotesi uscita dalla Commissione prevede una fattispecie che colpisce qualsiasi privato investito di una qualche funzione di professionalità, non meglio specificata. Delle due l'una: o ha sbagliato il Governo nel prevedere che la norma comunitaria potesse essere attuata con il testo approvato a suo tempo

da una figura criminale a un'altra completamente diversa, molto più ampia e sfumata, nella quale si possono inserire

perché vanno al di là di ogni possibile immaginazione sul piano dell'applicazione pratica. Allora, Presidente, l'accantonamento mi sembra necessario anche per chiarire questo punto di adesione del testo della Commissione al contenuto della decisione quadro citata nell'intitolazione dell'articolo, che è la stessa sia del vecchio articolo 19 che del nuovo articolo 31. Non è cambiato nulla, la decisione quadro è la stessa, però le due ipotesi sono completamente e radicalmente diverse. Chiedo un chiarimento sotto questo profilo e l'accantonamento mi sembrerebbe del tutto ragionevole.

non definita nei dettagli, scardina un principio del nostro ordinamento, ossia che i reati economici svolti tra privati siano procedibili per iniziativa di parte.

la procedibilità d'ufficio. Tutti riusciamo a capire che si tratta di contenere un fenomeno che concerne i dipendenti infedeli, ma sappiamo che vi è un contraltare della rigorosità con cui deve operare il funzionario pubblico. Quest'ultimo è soggetto a reati di questo genere se non segue

direttamente o tramite intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura ad una persona, per essa stessa o per un terzo, che svolga funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di un'entità del settore privato affinché essa compia o ometta un atto in violazione di un dovere»**.** Subito dopo si dice che il paragrafo 1 si applica alle attività professionali svolte nell'ambito di entità a scopo di lucro e senza scopo di lucro. lucro. Risulta chiaro che l'inclusione nell'ambito dei reati societari operata dalla prima bozza del Governo era errata.

sopprimere le parole «a statuto ordinario»; altrimenti, lo votiamo così com'è, dato che, di per sé, affronta un tema di principio che, in sede di ulteriori provvedimenti, può essere estensibile anche ad altre realtà delle autonomie locali.

quella dell'ordine del giorno era solo un'ipotesi legata al suo eventuale accoglimento; quindi residua l'emendamento

per cui non mi sento di accogliere la sua proposta e, anche per uno spirito di coerenza complessiva rispetto alla questione, annuncio il voto contrario personale e del mio Gruppo sull'emendamento, se venisse mantenuto.

che dovrebbero passare dalle Regioni allo Stato) da quella dell'argomento trattato nell'emendamento 5.0.60 (che riguarda la possibilità che le Regioni effettuino queste spese senza considerarle nel computo ai fini del Patto di stabilità).

la differenziazione tra Regioni a statuto ordinario e Regioni a statuto speciale e quindi mi adeguo alla discussione che è stata svolta in Commissione bilancio. Non chiedo una modifica del testo dell'emendamento, ma lo mantengo fermo perché, ripeto, sono due

verrà disatteso, come purtroppo accade al 99 per cento degli ordini del giorno, approvati dal Governo su indicazione di proponenti in questa Assemblea. Ripeto, qui si tratta di un emendamento che serve ad esentare le Regioni dal computo nell'ambito del Patto di stabilità di spese sostenute in materia ambientale per superare infrazioni comunitarie in campo ambientale. Credo sia assolutamente legittimo che le Regioni possano evitare il computo di tali spese nell'ambito del Patto di stabilità. Pertanto, mantengo l'emendamento e ne chiedo l'approvazione anche ai proponenti, che mi dispiace abbiano avuto un ripensamento sull'argomento.

l'emendamento viene ritirato per essere trasformato in ordine del giorno, viene preclusa la possibilità Ho seguito personalmente l'intervento del senatore Silvestri, il quale già nel suo intervento aveva preannunciato tale possibilità.

che ritengo assolutamente non congruente con la nostra discussione che l'emendamento del senatore Silvestri, che ho fatto mio, non sia stato posto in votazione.

Presidente, chiedo al Governo di accogliere il mio ordine del giorno che va nella direzione di mettere sullo stesso piano la sicurezza e la salute delle popolazioni che sono prossime a tutti i valichi alpini, quali il traforo del Monte Bianco ed altri, senza che talune siano privilegiate rispetto ad altre.

il significato e il contenuto dei due ordini del giorno e dell'emendamento che ho proposto, che sono frutto di un lavoro che abbiamo svolto in Commissione di approfondimento rispetto alle strategie, alle politiche delle istituzioni finanziarie internazionali, Banca mondiale, in primo luogo, che ci hanno portato a condividere con i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche con esponenti dei movimenti sociali e di ONG auditi, una serie di preoccupazioni e di di esortazioni che vorremmo appunto rivolgere al Governo attraverso questi due ordini del giorno. L'ordine del giorno G100 riguarda la Banca asiatica per lo sviluppo e si chiede di seguire la linea già intrapresa di maggiore coerenza e di efficacia nell'intervento della Banca asiatica per lo sviluppo, in particolare per quanto riguarda la lotta alla povertà e le strategie di sviluppo sostenibile e valutazione d'impatto ambientale e sociale dei progetti da essa finanziati. Quindi, riprende un ordine del giorno già approvato nella scorsa legislatura e lo fa proprio. Il G200 è un ordine del giorno sulla IAD, struttura della Banca mondiale che si occupa di lotta alla povertà. Chiediamo, anche sulla scorta della grave crisi di credibilità che la Banca ha attraversato e tuttora attraversa dopo lo scandalo che ha colpito l'allora presidente, Paul Wolfowitz, e anche per i ritardi di questa istituzione nel tener fede ai propri impegni di lotta alla povertà, di approvare questo ordine del giorno nel quale si chiede di sostenere una moratoria ai processi di privatizzazione dell'acqua e di riconoscere l'acqua come bene comune fondamentale, in linea con una mozione già approvata all'unanimità alla Camera. L'emendamento 11.0.200 amplia amplia un emendamento già approvato nella scorsa legislatura, chiedendo al Governo di rendere note le posizioni riportate dai nostri rappresentanti nelle banche multilaterali di sviluppo e di darci una valutazione di come queste istituzioni finanziarie contribuiscano al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nel millennio.

regolamentare o attraverso una decisione della Presidenza (specie in questo momento e per il caso specifico che mi permetterà di illustrare) che quantomeno l'ordine del giorno debba avere un contenuto proprio che possa essere riconducibile a quello dell'articolo a cui l'emendamento e l'ordine del giorno si riferiscono.

dà delega al Governo di introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, mentre l'ordine del giorno

scorso. Sulla stampa odierna, circa il disastro aereo di San Paolo in Brasile, leggo che il pilota non è riuscito a frenare perché non ha trovato davanti a sé, come in tutti gli aeroporti, un prato ma una strada congestionata dal traffico: su questa strada c'era una macchina con a bordo una mamma e la sua bambina trovate poi carbonizzate. Purtroppo l'accaduto è attinente alla mia interrogazione. Nell'aeroporto di Ciampino, con la Via dei Laghi ai margini della testata della pista, si potrebbe ripetere - mai ci auguriamo che accada - il disastro di San Paolo. basterebbe autorizzare la complanare alla Via dei Laghi progettata dal Comune di Ciampino. Purtroppo l'ignavia regna sovrana, in certi ambienti della pubblica amministrazione, al punto che sono passati ormai tre mesi

che è sotto gli occhi di tutti, però sarebbe bene fornisse le indicazioni che ho chiesto anche per una valutazione da parte degli storici su quella

Presidente, richiamo la sua attenzione sulle dichiarazioni di qualche giorno fa in Commissione affari costituzionali

del mio Gruppo me lo ha detto, quindi non ho motivo di dubitare del contrario, che sia stato distribuito ai Capigruppo il testo di riforma della previdenza dei senatori. Mi permetto di sollecitare lei, come Presidente dell'Assemblea di turno, perché venga rispettato l'impegno formale che così solennemente ha assunto il presidente Marini la settimana scorsa e non ho dubbi che da parte dell'intera Presidenza si voglia rispettare tale accordo. Mi permetto di sollecitare

della regolamentazione della previdenza dei senatori, nel Paese saranno poi tutti i senatori a rispondere del tipo di riforma che verrà adottata. Lei sa, Presidente, che c'è un documento redatto in forma di articolato, con relazione di accompagnamento, sottoscritto da 31 senatori, molti me lo hanno continuato a chiedere, lo hanno ricevuto in seconda lettura (intendendo significare che lo hanno ricevuto per la seconda volta), evidentemente c'è un interesse, non vorremmo che si rimanesse alle agenzie di stampa e agli articoli dei giornali senza avere di disporre del testo di articolato, che verrà in discussione nell'organo competente, prima della deliberazione. Ripeto, sarebbe importante che i parlamentari, in questo caso i senatori, ne potessero discutere in assemblea di Gruppo con i propri Presidenti e poi questi ultimi riferire,

quale, oralmente, è stata data informazione dei contenuti rispetto alle modifiche che si andranno ad approvare. Il testo scritto non l'ho visto, né mi risulta che esista allo stato dell'arte.

in vista di un prossimo Consiglio di Presidenza, sono certo e voglio augurarmi ci si arrivi con un esame accurato dell'articolato e non certo di un articolato che si trovi sul tavolo al momento del voto.

Signor Presidente, intervengo perché vorrei che lei sollecitasse il Presidente del Senato a sottoporre alla Giunta per il Regolamento alcuni accadimenti da me sottolineati da tempo in quest'Aula, perché stiamo perdendo un po', a mio giudizio, il filo di modi comportamentali che avevano, per la mia esperienza ormai quasi quindicennale, retto i lavori della nostra Assemblea. Mi riferisco ad una interpretazione corretta dell'articolo 76 in tema di riproponibilità dei disegni di legge già respinti, da me sollevato

da questa Assemblea nell'ottobre del 2006 e riproposto nel febbraio (quindi entro il termine dei sei mesi) e posto in discussione. Così come alcuni giorni fa

bisogna che si intervenga con una puntuale rilevazione di come ci dobbiamo comportare. Peraltro, quell'episodio di alcuni giorni fa non è dissimile da quello che si è verificato oggi, è stato ammesso un ordine del giorno che non aveva alcun riferimento con l'emendamento ritirato, che quindi non doveva essere dichiarato proponibile lasciando vivere l'emendamento in sostituzione del quale l'ordine del giorno era stato presentato. era stato presentato. Se dovessimo poter agire così, Presidente, significherebbe che in qualsiasi momento in quest'Aula si possono smontare e rimontare argomenti, trasformare e ritrasformare emendamenti, inserire nuovi emendamenti, trasformare emendamenti in ordini del giorno, con l'effetto di privare l'Assemblea della possibilità di discutere dell'argomento contenuto negli emendamenti perché sostituiti da ordini del giorno che con quegli emendamenti nulla hanno a che vedere. Ancor di più, l'ordine del giorno oggi ammesso in discussione e

da senatore che credo segua con una certa attenzione i lavori di questa Assemblea ormai da anni, con una discreta esperienza alle spalle, per il fatto che ci troviamo veramente nell'incertezza di come comportarci. Come ho detto, in questa incertezza molti ne profittano per cambiare